non ci sono gli emendamenti.

recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario***

si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 3, cioè quella norma che definiva l'ambito di sanatoria dei debiti pregressi dei produttori di latte. in Commissione bilancio abbiamo chiesto al Governo di chiarirci la portata normativa dell'innovazione proposta, perché da un lato sembrerebbe, sulla base del testo che ci è stato presentato, che la platea dei beneficiari della nuova disposizione si restringa, in quanto si prevede un'eccezione alla norma generale di rateizzazione (cioè quella riferita ai debitori per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea), dall'altro, però, scompare il riferimento ai produttori di latte. Se è così, così, ci chiedete - mi permetto di aggiungere - surrettiziamente e silenziosamente di introdurre una sanatoria di carattere generale riferita a tutti i produttori agricoli e non solo ai produttori di latte. In altri termini, anche i produttori di olio e non so quanti altri che ricevono provvidenze dall'Unione europea o sono soggetti a limitazioni da parte della stessa

il parere della Commissione bilancio risulterebbe palesemente viziato, giacché non si è tenuto conto, benché abbiamo espresso una contrarietà netta in quella sede, del potenziale enorme ampliamento della platea dei beneficiari. Infine, se così è, il Governo ci dica quanti e chi sono questi beneficiari e di quali importi stiamo discutendo, perché già ieri abbiamo sollevato un problema di enorme rilevanza, che non è stato risolto, relativamente al *quantum* di

senatore Morando

Per questo le chiedo di sospendere i lavori fintanto che il Governo su tutti i suoi emendamenti non avrà presentato la relazione tecnica. In secondo luogo, insisto sull'argomento appena sollevato dal senatore Legnini.

delle enormità tecniche e politiche contenute nella integrazione della relazione tecnica del Ministero dell'economia. Le garantisco che su quelle enormità torneremo a discutere in quest'Aula, perché si tratta di precedenti che hanno un rilievo istituzionale particolarmente importante.

gli articoli non si votano e quindi è sempre possibile tornare con un emendamento su un articolo le cui proposte di modifica sono già state discusse,

«pagando l'importo della rata annuale dopo aver rinunciato al contenzioso». contenzioso». Il ragioniere, che si rende conto che la parola giusta per questo provvedimento è condono, dice quindi: intanto aderisci al condono (mi scuso per la volgarizzazione) in quanto almeno

Esattamente questo: «accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso». La deflazione del contenzioso viene ora eliminata attraverso la presentazione di un emendamento del Governo che in sostanza fa venir meno le finalità fondamentali della norma.

Mi dispiace molto pronunciare queste parole, perché in tanti anni di attività, nella maggioranza o nell'opposizione, non le ho mai pronunciate: mi sono sempre fidato dei pareri tecnici del Ministero dell'economia, quale che fosse la mia collocazione, nella maggioranza o all'opposizione, e nessuno qui può smentire quello che sto dicendo. Mi sono sempre fidato, ma ora non lo farò più, perché il Ministero dell'economia questa mattina ci ha detto che l'emendamento 3.1000 restringerebbe la platea di beneficiari della cosiddetta rateizzazione.

che il presupposto su cui la Commissione bilancio ha deciso per il nulla osta questa mattina è tecnicamente inesistente. Questo emendamento amplia enormemente la platea dei beneficiari della rateizzazione, perché

l'ipotesi di intervento - e c'è da vedere pure su questo punto - ma è sicuro che la platea dei beneficiari della possibilità di rateizzare si amplia enormemente, andando molto al di là dei produttori lattiero-caseari. lattiero-caseari. Signor Presidente, a tutto c'è un limite. Mi sento ingannato dal Ministero dell'economia e le garantisco che non mi succederà più, non perché non tenteranno ancora di ingannarmi - cosa che è certa, per quello che mi riguarda - ma perché starò attento a non caderci, a differenza di quanto ho fatto questa mattina. Le dico un'altra cosa.

Napoli sono plateali e non hanno mai negato che fosse così e che si trattasse cioè di una porcata. Questa è una porcata che, per di più, ci viene proposta dai censori

Signor Presidente, colgo l'occasione per chiedere che sia consentito alla Commissione bilancio di lavorare. Questi inconvenienti possono capitare proprio per il continuo

orientamenti più disparati. Devo dire che il relatore questo lo fa, naturalmente, molto volentieri, perché è consapevole che su questo punto vi è una richiesta forte da parte di tutti i colleghi della Commissione agricoltura, che ho l'onore e il piacere di presiedere, e vi è una richiesta forte da parte di tutti i Gruppi politici, dimostrata in vario modo in tutte queste settimane. Vi è una richiesta altrettanto forte da parte di tutte, ma proprio tutte, le associazioni agricole del nostro Paese: voglio ricordare che Coldiretti, la più grande organizzazione agricola europea, e quindi anche italiana, e che rappresenta il 65 per cento dei produttori di latte, ha chiesto con forza che questo emendamento potesse essere inserito ed accolto. Dopo Coldiretti altre organizzazioni importanti, in particolare Confagricoltura e CIA, hanno fatto questa richiesta, anche organizzazioni di tutti gli orientamenti, comprese la Lega delle cooperative e la Confcooperative. Ritengo, quindi, che il fatto che oggi possa essere accolto questo

di ieri, noi avevamo presentato un emendamento analogo, il 4.11, su un punto che il Partito Democratico

Ieri abbiamo detto una cosa molto semplice: chi non ha rispettato la legge, prima di accedere a questa sanatoria, pagare gli arretrati e rinunciare ai contenziosi giudiziari che hanno bloccato il recupero delle multe passate. Ci sembra questo il punto di partenza per una battaglia per la legalità, che abbiamo ricordato ieri, perché non vengano premiati come al solito i più furbi e si stabilisca un principio di equità e giustizia per tutti gli allevatori seri che si sono indebitati per pagare le multe

un tentativo di mettere in parallelo due procedure che rischiano di andare ognuna per proprio conto: una relativa al recupero delle multe e l'altra relativa all'assegnazione delle nuove quote. Ci piace immaginare che ci sia una garanzia nei confronti dello Stato che si sta spendendo per ricostruire un sistema di reingresso per coloro che non hanno rispettato le regole. dà la possibilità all'AGEA, che gestisce le risorse, di trattenere in via anticipata le quote delle rate non ancora versate a garanzia dei successivi pagamenti da parte degli splafonatori. Questo aumenterebbe il livello di sicurezza rispetto ad una apertura di credito nei confronti di coloro che in questi ambiti hanno dimostrato di essere un po' refrattari.

giunta ieri la comunicazione con cui si introduce un nuovo principio, che immagino verrà adottato anche nelle prossime occasioni, visto e considerato che la normativa vigente in materia tributaria

Signor Presidente, intervengo per chiederle una correzione del resoconto della seduta pubblica di ieri, perché, come risulta nell'originario fascicolo degli emendamenti, stampato e distribuito in Aula, all'emendamento 6.0.4, recante proroga di agevolazioni previdenziali per le imprese agricole in zone svantaggiate, risultano apposte anche le firme dei senatori del Gruppo del Partito Democratico della Commissione agricoltura. Poiché lo stesso è stato successivamente riformulato, per un mero refuso, non risultano tutte le firme originariamente apposte, che invece, come tali, devono essere considerate. Del resto, correttamente, lo stesso relatore, Presidente della Commissione, senatore Scarpa Bonazza Buora, durante il suo intervento ieri in Aula, ha ritirato l'emendamento 6.0.3 della Commissione, stante il parere favorevole sull'emendamento 6.0.4 6.0.4 (testo 2), presentato da numerosi senatori di maggioranza e di opposizione, che fa propria la sostanza dell'emendamento precedente della Commissione agricoltura, recante la proroga delle agevolazioni contributive fino al 31 dicembre dicembre di quest'anno. Una richiesta, tra l'altro, più volte avanzata dal Gruppo del Partito Democratico in Commissione agricoltura, in vari provvedimenti, dalla finanziaria al decreto competitività, dal decreto anticrisi al cosiddetto decreto milleproroghe. Una richiesta più volte più volte avanzata e più volte rigettata dal Governo e che oggi trova nel decreto sulle quote latte parziale accoglimento, avendo l'Esecutivo rigettato la proposta del Gruppo del Partito Democratico, di proroga

in modo particolare dal nostro Ministro, Luca Zaia, che, a nome di tutto il Gruppo, vogliamo comunque ringraziare per quanto ha fatto per l'intero settore in Europa, dove ha ottenuto importanti successi, a nostro modesto parere,

onorevoli colleghi, la rinuncia al contenzioso di chi vorrà aderire alla rateizzazione delle multe è un principio importante, che viene riconosciuto. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi successivi.

Tutti noi della maggioranza - perché siamo una maggioranza, collega Bodega, non siamo solo un Gruppo, non siete solo un Gruppo: siamo una maggioranza che sostiene un Governo e che sostiene un Ministro

la disciplina della produzione nazionale di latte e la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, è senza dubbio importante. Tuttavia, a mio parere, pur condividendo l'improrogabilità di disciplinare tale materia, non ravvedo la necessità della decretazione d'urgenza, visto che la questione delle quote latte si trascina da 25 anni. Sarebbe stato più logico, invece, dare al Parlamento la possibilità di esaminare un provvedimento, non un decreto, al fine di ripristinare un maggiore un maggiore senso di giustizia e di garantire una prospettiva al settore zootecnico già fortemente provato da un mercato non favorevole. favorevole. Come ho già accennato nel mio precedente intervento - e pertanto non mi ripeto in questa sede - la Commissione agricoltura ha approvato alcune modifiche al testo originario, che sono ampiamente condivise da me e dal mio Gruppo. Al di fuori di tali disposizioni condivisibili, il decreto-legge in esame presenta un complesso di interventi in favore di coloro che fino ad oggi hanno operato al di fuori delle norme, e risulta essere un provvedimento discriminatorio nei confronti della grande maggioranza degli allevatori che, con enormi sacrifici, in questi anni hanno rispettato le regole. Il provvedimento prevede che le quote aggiuntive vengono assegnate soprattutto ai grandi splafonatori. Questi, infatti, saranno i soggetti privilegiati nell'assegnazione delle quote aggiuntive e non saranno tenuti neppure a rinunciare al contenzioso aperto contro lo Stato per temporeggiare sul pagamento delle multe. Così facendo, vengono messi in coda coloro che hanno pagato per avere le quote necessarie in affitto, limitando la restituzione della quota B tagliata al solo quantitativo prodotto in esubero, mentre i piccoli splafonatori vengono addirittura esclusi totalmente dall'assegnazione. In definitiva, il decreto che doveva regolamentare l'assegnazione di nuove quote, che dovrebbero essere disponibili dalla prossima campagna di aprile, contiene un vero e proprio *cadeau* per chi ha operato fuori dalle regole e viene riammesso, nonostante la legge nazionale, al meccanismo della compensazione, avvantaggiandosi di una riduzione sulle eventuali multe e a svantaggio ancora una volta di chi ha operato nella legalità. Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto contrario del mio Gruppo. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, due sono, in sostanza, le parti essenziali di questo decreto-legge: quella rivolta alla sistemazione delle posizioni e quella dedicata all'attribuzione di quota. Per quanto concerne la regolarizzazione delle posizioni, trovo legittimo che, da parte degli allevatori che con sacrifici e grandi esborsi hanno finora operato nel rispetto della legge,

che, nonostante le buone intenzioni dichiarate dal Ministro all'inizio dell'*iter* del provvedimento, si è invece dimostrato sordo a qualsiasi ipotesi migliorativa del testo proposta dall'opposizione. Ogni ulteriore concessione in tal senso sarebbe una scorrettezza nei confronti dei numerosissimi allevatori che hanno agito nella legalità. Per quanto riguarda, invece, i criteri di attribuzione delle nuove quote, anche in questo caso ci poniamo degli interrogativi. Siamo in presenza di una legge vincente, la n. 119 del 2003, che il Ministro non disconosce ma che di fatto, in questo caso, viene messa da parte per l'assegnazione delle quote. Ci è sembrato naturale, quindi, chiedere dei correttivi del testo in riferimento a tutti quegli aspetti del decreto che non premiano i produttori che in questi anni si sono mossi nel pieno rispetto della citata Faccio un altro esempio: sempre a proposito dell'attribuzione di quota, non ci sembra equo attribuire quota solo a chi ha prodotto quota B o la ha affittata senza tener conto di altre aziende che, sempre nel rispetto della legge e della legalità ma nel rispetto soprattutto degli allevatori che insieme a loro vanno avanti con grandissimi sacrifici, hanno compiuto la scelta di non utilizzarla. Noi che facciamo? Invece di premiarli, li danneggiamo,

Tra le proposte dell'Italia dei Valori, ricordo in particolare, la richiesta di modifica del decreto-legge finalizzata a fare in modo che gli allevatori che aderiscono alla rateizzazione debbano rinunciare ai contenziosi giudiziari. Ciò sarebbe stato

chiesto di abrogare la franchigia del 5 per cento della quantità splafonata, in quanto non sembra equo non considerare chi si è impegnato a mantenere il proprio aumento di quota nei limiti fisiologici, modificando altresì l'attuale meccanismo di rateizzazione, introducendo una norma che prevedeva che l'assegnazione di nuova quota facesse partire il pagamento del debito in modo tempestivo. Abbiamo chiesto altresì l'abrogazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1, la quale prevede, già nella campagna in corso, cioè in modo retroattivo, la restituzione del prelievo pagato in eccesso anche ai produttori non titolari di quota ed a quelli che hanno superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. Dobbiamo, purtroppo, registrare con rammarico che il Governo non ha tenuto fede alle promesse di modifica del testo al nostro esame. Infatti, il decreto-legge sulle quote latte non è stato modificato nelle sue parti più controverse, così come anche il Gruppo Italia dei Valori ha richiesto, insieme alle associazioni di categoria, soprattutto al fine di non vedere vanificati l'impegno e gli sforzi del mondo produttivo nel perseguire l'applicazione della legge n. 119 del 2003, votata da tutti i partiti, e per garantire i produttori che hanno sempre rispettato le regole. Voglio, inoltre, sottolineare che, proprio in questi giorni in cui si parla molto di federalismo, quindi di grande considerazione delle Regioni e degli enti locali, il ministro Zaia, espressione del partito che più degli altri preme sull'acceleratore di questa riforma, ha di fatto ignorato le Regioni, ha completamente cancellato la concertazione, varando un decreto-legge che riguarda solo una parte. L'agricoltura, così come denunciato dai tanti operatori del settore e da tutte le organizzazioni professionali di categoria, sta vivendo una fase drammatica, sicuramente la più acuta degli ultimi anni. Il Ministro fa finta di non vedere e non sentire e, mentre tutto il mondo dell'agricoltura chiede aiuti per cercare di frenare una crisi senza precedenti, vara un provvedimento che punta esclusivamente a salvaguardare i pochi "furbetti" che certamente non fanno gli interessi generali de! comparto. Il decreto-legge in esame, rappresenta un vero e proprio trattamento di favore per "gli irriducibili" "gli irriducibili" delle quote latte che hanno fino ad oggi operato al di fuori delle norme e nel pieno dell'illegalità. troviamo di fronte un provvedimento discriminatorio nei confronti della grande maggioranza degli allevatori che, con enormi sacrifici in questi anni, hanno rispettato le regole. Per questo, il Gruppo Italia dei Valori voterà contro questo decreto-legge, che ritiene inaccettabile, discriminatorio e assolutamente inadeguato a fare fronte alle reali esigenze degli operatori del settore lattiero-caseario. Vorrei infine rivolgere l'auspicio, con riferimento alle notizie pubblicate in questi giorni circa l'indagine della procura della Repubblica di Milano su presunti illeciti penali relativi al mancato versamento del prelievo sulle quote latte, latte, che l'indagine della magistratura possa fare chiarezza su una situazione che vede ormai da molti anni diffuse irregolarità, distorsione del mercato, nonché pregiudizio per i consumatori e per la grande maggioranza delle imprese produttrici. L'auspicio del Gruppo Italia dei Valori è che tutti gli operatori siano posti finalmente in un regime di uguaglianza e di giustizia, che vengano risarciti gli ingenti danni causati allo Stato si parla di oltre 90 milioni di euro - e che venga fatta giustizia nei confronti di chi è stato leso dai gravi illeciti commessi nell'ambito del sistema di frode ideato per eludere la normativa sulle quote latte.

dividendo il mondo agricolo e dando vita ad un contenzioso giuridico veramente notevole. Oggi stiamo parlando di oltre 8.400 aziende che rischiano di chiudere.

A suo tempo l'obiettivo era quello di garantire un valore al prezzo del latte, limitandone la quantità prodotta. L'intenzione, quindi, era buona: si cercava di sostenere il prezzo sui sui mercati contenendo la produzione. Peccato poi che, in sede di trattazione e di mediazioni a Bruxelles, si sia svenduta - e sottolineo svenduta - la nostra agricoltura, la nostra capacità produttiva, quindi la forza dei nostri agricoltori. Oggi, abbiamo la possibilità di produrre appena metà del latte che consumiamo; ritengo quindi sia umanamente comprensibile produrre di più rispetto a quanto la Comunità europea ci aveva riconosciuto, nonché giustificabile,

lo fa utilizzando i risultati notevoli - su questo siamo tutti quanti d'accordo - ottenuti dal ministro Zaia in sede di trattativa europea a Bruxelles. È evidente che, se noi oggi siamo qui a ragionare e discutiamo su questo argomento, è perché finalmente qualcuno si è messo a lavorare intensamente, è andato a Bruxelles e ha portato a casa dei risultati, altrimenti oggi non saremmo qua. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Si è ottenuto di poter usufruire di un aumento di 620.000 tonnellate, pari al 5 per cento della quota di produzione, da utilizzare *cash*, subito. Questo è un grande successo per noi, per il nostro Paese, per poter aiutare gli allevatori a uscire dalla illegalità generata da un sistema ingiusto, che andava gestito meglio allora, in tutt'altro modo, un sistema certamente non voluto dalla Lega Nord, che è sempre stata - e oggi lo sta dimostrando ancora più di ieri - vicina al mondo degli agricoltori. Oggi, grazie all'accordo di revisione della PAC, diamo la possibilità alle aziende rimaste fuori dalla legalità di rimediare non attraverso una sanatoria, ma con un'operazione di rientro finanziario.

Chi oggi parla di sanatoria, di illegalità e di ingiustizia forse dimentica - e credo, anzi spero, si tratti solo di poca memoria da parte di quelle persone - che l'ex ministro De Castro durante il Governo Prodi fece un condono previdenziale sui contributi SCAU di cui beneficiarono solo ristrette aree del nostro Paese, e lo fece, tra l'altro, con un atto amministrativo che non è neanche transitato per il Parlamento. sanatoria, allora sì, andava bene; oggi la rateizzazione del debito no, non va bene.

al nostro esame chi vuole entrare nella legalità può farlo tranquillamente, attraverso un percorso economico a tassi di interesse di mercato. Credo che il 6,5 per cento, che è il tasso di riferimento della Commissione europea, sia più che giusto, visti i tempi che corrono prevede il decreto, viene scaglionato in relazione all'importo e alla durata della rateizzazione. Chi si impegna oggi a rateizzare paga sicuramente di più di chi lo ha fatto in passato; è ingiusto, quindi, e sicuramente politicamente scorretto, parlare oggi di una sanatoria. In tutto questo, va sicuramente sottolineato e riconosciuto il coraggio del Ministro e del Governo nel volere affrontare temi che da venticinque anni sono lì, triti e ritriti, e che mai nessuno è riuscito a risolvere. Temi sui quali tutti quanti i Governi si sono adoperati per cercare rimedi, ma nessuno ci è riuscito fino in fondo. Credo sia notevole l'impegno sul lavoro profuso, tutti quanti abbiamo cercato di trovare la quadratura della questione, lavorando sicuramente sicuramente in maniera trasversale: il Ministro, il Governo e la Commissione agricoltura hanno sempre cercato costantemente e continuamente di risolvere in maniera costruttiva il problema. Il decreto, nella sostanza, mira a trovare una soluzione positiva, positiva, risolvendo contenziosi di chi ha prodotto in eccesso, non dimenticando, però, e, anzi, rispettando e dando una mano a chi è già in regola e si è da tempo immesso nel circuito della legalità. Non ci siamo certamente dimenticati di chi in passato

Credo vada inconfutabilmente dato atto al Ministro di aver fatto tutto il possibile su tale questione. Va ringraziata la Commissione agricoltura, presieduta

Non possiamo noi politici - mi rivolgo soprattutto agli amici di centrosinistra - contribuire ad innescare delle guerre tra poveri. Dobbiamo unirci ed essere compatti e solidali per affrontare le sfide del mercato, recuperando le molte occasioni che in passato, purtroppo, non per colpa della Lega, sono state perse in questo settore. Dobbiamo rendere l'impresa agricola il centro di gravità del sistema economico, creare un nuovo patto tra consumatori e produttori, difendere il consumatore da ogni forma di pirateria alimentare, valorizzare quanto più possibile qualità e territorialità dei nostri agricoltori, usando l'unico modo possibile per risolvere le sorti e rendere competitive tutte le aree del nostro Paese. L'unico modo è il federalismo, unico vero collante del nostro Paese. Solo con il federalismo, valorizzando ed incentivando le peculiarità dei vari territori, le tipicità locali e tutte le positività con la forza delle varie aree geografiche,

la forza dell'agricoltura del nostro Paese. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quella delle quote latte è certamente una questione da chiudere. Noi siamo d'accordo: è questione annosa e dannosa per questo Paese; è zavorra che va tolta dai tavoli europei e dalle trattative internazionali, perché ci vincola e penalizza. Siamo d'accordo con il Ministro. È, soprattutto, un singolare ed anomalo buco nelle casse dello Stato che pesa sulle spalle dei cittadini, una mancata disponibilità finanziaria per oltre un miliardo e mezzo non è solo una questione di settore, ma incrocia diritti di tutti e ingiustizie diffuse. Allora, per noi, chiuderla, ancora di più, vuol dire chiuderla bene e in controtendenza rispetto a ciò che è stato fin qui. Non vuol dire perpetuare iniquità, non a prescindere, come è stato ben detto da una mia collega, ma voltando pagina. Questo abbiamo detto al ministro Zaia sin dall'inizio, quando ci ha delineato il profilo e l'impostazione del decreto. Abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare lealmente, costruttivamente, a condizione che il provvedimento contenesse i punti fondamentali, che fosse caratterizzato come il decreto che pensa e riparte da chi ha onestamente faticato per riequilibrare la propria produzione, riportandola nell'ambito delle regole. Lo hanno sostenuto bene e puntualmente i miei colleghi del Gruppo PD e della Commissione agricoltura, oltre punto sta nell'ordine di assegnazione delle quote. Noi abbiamo detto che, senza dubbio alcuno, le quote vanno prima assegnate a chi ha pagato, a chi si è indebitato per mettersi in regola, a chi ha impegnato le stesse quote come garanzia, non avendo altro da impegnare; sarebbe data priorità a chi ha affittato, cercando anche forme diverse ma comunque onerose per regolarizzarsi, non mescolando affittuari e splafonatori, come rimane stabilito In sostanza, prima tutti coloro che hanno fatto sforzi veri e che, mentre si accollavano oneri anche pesanti, anche a rischio della tenuta delle stesse aziende, dovevano competere in un mercato viziato, alterato da latte in nero, fuori quota, fuori da ogni regola, così dal 1984. In questo modo, per anni, si è operato in una concorrenza più che sleale tra imprenditori in regola e chi continuava imperterrito a produrre oltre il 100 per cento delle proprie quote, nonché con chi continuava a produrre addirittura senza quota alcuna. E non stiamo parlando - si badi bene - di piccole aziende o di agricoltura di sussistenza. Due dati bastano a dimostrarlo: se sono 606.000 le tonnellate di latte prodotte fuori quota in Italia, 450.000 tonnellate sono state prodotte dai grandi splafonatori, ovvero il 75 per cento dello splafonamento nazionale è dovuto alla produzione in eccedenza dei supersplafonatori. Sono molte aziende? No, sono l'1,58 per cento. L'1,58 per cento ha prodotto il 75 per cento del fuori quota italiano. Ecco il perché della rabbia che sta uscendo nelle piazze, nelle assemblee, il perché di quelle migliaia di firme raccolte in un sol giorno in Lombardia. richiesta di giustizia e trasparenza alla fine di un lungo percorso durato anni che giusto non è stato, equo non è stato. È una richiesta volta a che oggi questo provvedimento sia, finalmente, un atto che spinga a comportamenti etici,

Chiamiamola condono: è lo stesso. Ma se condono deve essere per non far chiudere quelle aziende - e noi non vogliamo far chiudere nessuno, tanto meno in agricoltura, tanto meno ora, nel mezzo di una crisi colossale colossale - sia fatto con serietà e rigore, a partire dai presupposti che lo sorreggono, dalle coperture finanziarie, perché sia possibile davvero la rateizzazione. Sia definito un percorso chiaro, credibile, che si paghi davvero, che siano rateizzazioni in tempi minimamente congrui e verificabili, che non venga assegnato nulla se non è stato avviato il percorso di pagamento. Soprattutto, abbiamo detto dal primo giorno, mettendolo per iscritto, chi ha aperto azioni legali e contenziosi avrebbe dovuto ritirarli. Ma in quale Paese del mondo, signor Ministro, lo Stato fa un patto con gli imprenditori, condona, concede, riammette ciò che era inammissibile, illegale,

Noi oggi siamo contenti del fatto che la Commissione bilancio ed il Ragioniere generale dello Stato abbiano confermato ciò che abbiamo sempre sostenuto con una logica semplice e lineare: o si fa un patto tra galantuomini o si va allo scontro in tribunale. Le due cose in contemporanea non possono stare. *(Applausi dal Gruppo PD).* Infatti, allora non più di patto si tratta, ma è l'ambiguità, è l'aggiustamento di volta in volta, è ancora l'Italia delle furberie se si può, dei rinvii e poi qualcuno provvederà. Noi ne abbiamo fatto un punto centrale delle nostre condizioni, ma devo dire che non abbiamo inventato nulla. Leggo un passaggio di una lettera scritta ad un allevatore dal Ministero nel 2003: «Per poter usufruire della rateizzazione è necessario mettersi in regola, provvedendo subito a versare il prelievo supplementare relativo all'ultima campagna 2002-2003 e rinunciare espressamente a qualsiasi contenzioso legale pendente per tutte le campagne trascorse». Firmato: ministro Alemanno. Ora finalmente, con il parere della Commissione bilancio, tradotto e trasmesso all'Aula dal relatore, viene ripristinato il punto fondamentale, il senso di giustizia; avremmo preferito, signor Ministro, che lei fosse davanti in quest'impostazione e non a rimorchio, non con la fragile giustificazione, che abbiamo sentito ripetere questa mattina, che ci sono differenze tra quella campagna ed ora, determinate dagli interessi che in questa rateizzazione sono presenti. Noi rimaniamo con la sensazione che lei l'abbia subito e crediamo anche che abbia perso una grande occasione per fare un patto vero con gli imprenditori. Abbiamo chiesto, inoltre, con forza l'istituzione di un fondo effettivo, dedicato subito al sostegno delle imprese oneste e virtuose, un fondo ora e non poi, se qualcosa avanza dopo il recupero dei debiti. Abbiamo chiesto 500 milioni dedicati, gli stessi che lei, signor Ministro, aveva promesso con il primo annuncio di questa operazione. I 500 milioni sono diventati 25, poi 35 in un emendamento, poi bocciati dalla 5a Commissione perché non coperti, poi riapparsi in serata *in extremis*, che sottrae 20 milioni ai piani di settore forestali, un altro danno creato per coprire un danno preesistente. Credo che l'istituzione di un fondo coperto con risorse certe, considerato priorità vera di questo Governo, avrebbe avuto da solo una forza di portata dirompente, sia sul piano economico, sia sul piano etico. Sarebbe stato un messaggio forte tale da far pensare ai giovani imprenditori che, allora, stare nelle regole conviene; che non è la stessa cosa seguire la legalità o non farlo. Sarebbe stato un segnale di riconoscimento non solo per lo sforzo fatto, ma per l'apertura di un nuovo tempo che si lasci alle spalle l'Italia degli *escamotage*. Noi non diciamo no anche ad un solo euro messo in agricoltura, che possa essere utile ad innovare, a crescere e non solo ad assistere, ma non ci stancheremo di dire che è ora di programmi e non di *boutades* e di improvvisazioni. È una vergogna che il fondo per le garanzie assicurative oggi, ancora una volta, trovi zero risorse; risorse che già c'erano, che servivano a far fronte alle calamità climatiche in crescita, che mettono in difficoltà centinaia di aziende. La verità è che si fanno grande azioni comunicative, ma non si prevede neppure ciò che c'era e che serve. Sulle agevolazioni previdenziali per le zone svantaggiate, che sono il Sud e il 50 per cento dell'Italia fatto di montagna, noi abbiamo aderito agli emendamenti *bipartisan* della Commissione e all'emendamento approvato in Aula, ma abbiamo anche riproposto, attraverso i nostri emendamenti, l'urgenza che vengano fatti programmi pluriennali. Quale impresa può fare programmi, piani industriali di tre mesi in tre mesi, di settimana e in settimana? È, ancora una volta, la spinta all'improvvisazione, all'arrangiarsi: nessuna cultura dell'imprenditorialità si costruisce così; quella che, invece, servirebbe, la prima cosa che serve al sistema agricolo italiano, che per salvarsi deve internazionalizzarsi, deve competere, deve ricercare e ha bisogno di tempi lunghi per questo. Bene, lei, signor Ministro, ha introdotto qualche cambiamento, mezzo cambiamento, ha accolto i nostri emendamenti, pochi per la verità e non quelli sostanziali, che comunque hanno concorso a mitigare i paradossi che erano presenti nel testo originario. Altri ci pare li abbia subiti, come quello sui contenziosi, ma una cosa è certa: questo provvedimento uscirà dal Senato diverso da come è entrato e noi siamo contenti di avere concorso a modificarlo. Noi le riconosciamo di essersi impegnato nella mediazione, ma il problema è che non ha avuto il coraggio di apportare una inversione di tendenza vera e di cambiarne il tratto, o meglio ha svolto un ruolo da amministratore delegato degli agricoltori, come lei si definisce. Ma questa volta non basta: serve la politica, quella con la P maiuscola, che sulla bilancia non metta solo le entrate, le uscite, le mediazioni e i contratti, ma usa concetti come etica, principi, orgoglio dei valori, quelli che stanno fuori dalle contrattazioni, perché non sono contrattabili. È questo che le stanno chiedendo dalle piazze e di cui lei sembra addirittura sorprendersi. Ma ciò che stride di più, lasciatecelo dire, è che questo provvedimento viene proposto da un Ministro che appartiene ad un partito, la Lega Nord, che mentre predica il federalismo, come anche poco fa il collega Vallardi, qui toglie alle Regioni le competenze che avevano. Mentre fa della legalità la sua bandiera e dal Nord impartisce grandi lezioni sulla legalità a Napoli e dintorni, qui si defila in sordina facendo finta che di legalità non si tratti. Stride che Alleanza Nazionale abbia deciso di mettere via e di rinnegare la legge n. 119 del ministro Alemanno che, nel momento più difficile ed acuto del problema delle quote latte, ha saputo tenere ferma la barra e promuovere responsabilmente un sistema basato su presupposti di rigore e legalità, come si è letto nella lettera citata. Noi quella legge la votammo. Noi abbiamo cambiato nome nel frattempo, ma quei princìpi sono rimasti saldi dentro di noi. Noi siamo coerentemente su quelle posizioni. Noi diciamo convintamente al mondo dell'agricoltura che anche dalle crisi più pesanti bisogna uscirne, sì, insieme, ma con patti trasparenti, costruiti su presupposti di equità e giustizia. Questo provvedimento non dice questo. Non ci rappresenta e per tale motivo esprimiamo convintamente voto contrario.

il provvedimento che ci apprestiamo a votare, ribattezzato da tutti «decreto quote latte», segna - ed era ora - l'epilogo di una angosciante vicenda che si trascina ormai da venticinque anni e che, solo nell'ultima campagna lattiera, è costata all'Italia 160 milioni di euro di euro di multe, con 2 miliardi e mezzo di euro già versati negli anni alla Comunità europea. Sono numeri che evidenziano, se ancora ve ne fosse bisogno, una situazione inaccettabile. Una situazione nata nel 1984, quando, per far fronte alle rilevanti eccedenze di latte e suoi derivati si decise, in sede di Comunità europea, di regolarne la produzione, quando l'allora Governo - ed in modo particolare il Ministro dell'agricoltura - presero per buono un dato sulla produzione italiana che, nella sua determinazione, nascondeva quell'errore che, da allora, ha gravemente penalizzato il settore lattiero-caseario italiano e, in generale, la nostra economia. Un errore madornale che assegnò all'Italia quote latte per una quantità di gran lunga inferiore alla produzione e al consumo nazionale. Un errore madornale che induce al sospetto che, allora, qualcuno abbia "svenduto" l'agricoltura italiana, che non l'abbia saputa o voluta difendere. Uno sbaglio o una volontà politica che si è tradotta, negli anni, in un danno enorme per il sistema Paese. Uno sbaglio o una volontà politica che ha consentito che in Italia si consolidasse un mercato parallelo per il latte, per soddisfare una richiesta interna di materia prima, e che ha istituzionalizzato di fatto la nostra condizione di Paese importatore. Come era evidente, infatti, negli anni successivi al fatidico 1984, la produzione italiana di latte sforò oltre il tetto imposto dalle quote, in grado di coprire appena il 50 per cento del fabbisogno nazionale, e scattò il famigerato meccanismo sanzionatorio. Dapprima fu lo Stato, anziché i singoli produttori, a pagare milioni di euro alla Comunità europea, poi, con il pronunciamento della Corte di giustizia europea fu imposto il pagamento delle multe direttamente agli allevatori. E da qui l'apertura di numerosi contenziosi giudiziari e di altrettante sospensive concesse dal Tribunale amministrativo regionale; da qui la situazione di difficoltà di numerose aziende italiane travolte dai debiti; da qui il perdurare di una situazione insostenibile per lo Stato, per gli allevatori e per la zootecnia italiana. Un danno in molti casi irreversibile per tutto il sistema Paese. Oggi, colleghi - dobbiamo darne atto - questo Governo e il ministro Zaia in particolare hanno avuto il coraggio e la determinazione di affrontare il problema, prospettando una serie di interventi destinati a riporre definitivamente nel cassetto quella mannaia che per venticinque anni ha gravato su migliaia di aziende italiane, ad iniziare dall'eccellente lavoro che, con l'autorevolezza del presidente Berlusconi, ha consentito all'Italia di riacquistare in sede europea quella considerazione, quel prestigio e quel rispetto che, da troppo tempo, mancava al nostro Paese. Non dimentichiamoci, infatti, che questo decreto arriva subito dopo l'accordo con Bruxelles, siglato il 20 novembre scorso, e che ha attribuito all'Italia 620.000 tonnellate di produzione in più. Non dimentichiamoci che i contenuti di questo decreto rappresentano una proposta concreta ai problemi derivanti dalla sovrapproduzione lattiera, una proposta concreta contrapposta alla latitanza di chi in passato, pur avendone titolo, ha preferito non occuparsene e che, oggi, magari cavalca e strumentalizza qualche malumore, fuori e dentro quest'Aula. Noi del PdL siamo coscienti che sia difficile accontentare tutti, così come è difficile predisporre un testo in grado di trovare la difficile sintesi tra le esigenze di quanti si sono sempre attenuti al rispetto dei limiti e quanti oggi vengono messi in condizione di farlo, tra le restrizioni imposte dalla Comunità europea ed il fabbisogno nazionale, tra le multe da pagare ed il rischio fallimento di molte aziende italiane. Ma è evidente, e non devo convincere nessuno, abbiamo davanti un provvedimento equilibrato, frutto di una azione mediata, svincolato dalle *lobby* nostrane ed europee, un testo ben ragionato, che non si fa condizionare da interessi diversi, se non quelli dell'agricoltura italiana. Un testo sicuramente perfezionabile nel percorso parlamentare. Colleghi, questo, non lo era in Commissione e non è oggi in Aula un testo blindato, non lo è mai stato per espressa volontà del ministro Zaia, come confermano le numerose audizioni, formali ed informali, dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del mondo delle cooperative. Questo non è un decreto che premia i furbi, come qualcuno vuol far credere, ma non lascia neanche spazio ai furbi, a coloro i quali, per interessi diversi e personali, vogliono speculare sulle spalle degli allevatori. Colleghi, ammiro chi all'interno del mondo agricolo organizzato si fa carico di risolvere il problema e di concertare gli interventi a solo vantaggio dell'agricoltura italiana e rispetto anche la protesta degli allevatori, in buona fede. Apprezzo poco o niente, invece, le devianze di alcuni dirigenti, che sono più attenti alla scalata alla poltrona di qualche presidenza che non a difendere la nostra agricoltura. Invece di orientare i trattori verso le residenze private del presidente Berlusconi e del ministro Bossi, perché non si sono preoccupati di orientarli, in questi anni, verso chi ha causato il problema e, soprattutto, verso chi non ha fatto nulla per risolverlo? *(Applausi dal le posizioni di chi utilizza il decreto sulle quote latte per portare avanti la sua piccola e privata guerra personale, di chi usa le organizzazioni per la sua azione ideologica, di chi, invece di occuparsi degli interessi degli allevatori, fa politica all'interno delle organizzazioni agricole. E da allevatore, mi rivolgo agli allevatori: attenti a non farvi strumentalizzare da personaggi interessati esclusivamente al proprio tornaconto personale! In questo momento serve a poco prestare il fianco a chi fomenta la protesta, cieco rispetto al male che sta facendo all'agricoltura ed al Paese. Smettiamola con le azioni demagogiche, diamo il merito al Governo Berlusconi ed al ministro Zaia di aver fatto finalmente tornare l'Italia protagonista in una trattativa comunitaria e, soprattutto, di aver individuato una soluzione ad una vicenda che per gli allevatori, per il Paese, e per tutti noi rappresentava un danno economico e di immagine senza eguali. Colleghi, ora guardiamo oltre, c'è bisogno di guardare oltre. Siamo tutti coscienti che questo settore primario e strategico va difeso e sostenuto: lo è l'Europa, lo sono il presidente Berlusconi e il ministro Zaia e mi auguro che lo siano i colleghi della minoranza. Noi del Popolo della Libertà sappiamo che occorre uno impegno concreto per far tornare l'agricoltura il cuore pulsante dell'economia del Paese. E lanciamo una sfida, una sfida che prevede un progetto agricolo italiano, un piano strategico, in parte già avviato, che possa dare agli imprenditori agricoli un futuro fatto di maggiori certezze. Infatti, colleghi, la nostra agricoltura è qualità, è eccellenza alimentare, è motore dell'*export*, è volano di nuove economie. Certo, serve di più. Serve un'adeguata tutela commerciale del prodotto zootecnico. Serve sconfiggere il fenomeno del latte in nero. Serve assicurare la tracciabilità e la qualità delle nostre produzioni. Serve una maggiore tutela del prodotto *made in Italy*. Serve combattere la pirateria agroalimentare. Serve assicurare gli agricoltori dai rischi connessi alla loro attività (e quindi, durante l'*iter* parlamentare, bisogna trovare le risorse). Serve la proroga della fiscalizzazione degli oneri contributivi per le aree montane e svantaggiate. Serve difendere l'agricoltura. Ma, soprattutto, serve dare ossigeno ad un'agricoltura sempre più morente. E questo provvedimento, colleghi, così come gli altri interventi del ministro Zaia, va in questa direzione. Il mondo, l'Europa e l'Italia, travolti da una crisi senza precedenti, riconoscono all'unisono il ruolo strategico e primario dell'agricoltura. Un'agricoltura che nel nostro Paese, con le sue 1.700.000 aziende, produce un valore aggiunto di 26 miliardi e contribuisce per oltre il 2 per cento al prodotto interno lordo. Un'agricoltura che però deve riacquistare la sua dimensione e il suo ruolo, per continuare ad essere protagonista attiva e per fornire il suo insostituibile contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese. Sono convinto - e concludo, signor Presidente - che il Popolo della Libertà, il Governo Berlusconi e il ministro Zaia abbiano la volontà, la competenza e la determinazione per occuparsi di tutte le esigenze del mondo agricolo. Ne è testimonianza non solo questo provvedimento, ma anche il disegno di legge per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare. La sfida è su questo piano, colleghi della minoranza. Basta con le inesattezze, basta con le devianti visioni che aumentano il senso di smarrimento degli agricoltori e danneggiano non solo l'agricoltura italiana, ma tutto il sistema Paese. Se realmente auspicate un mondo agricolo sano, competitivo e moderno, lasciate questo atteggiamento che favorisce lo scontro tra poveri e fatevi carico della responsabilità di contribuire a risolvere i problemi. Ministro, noi del Popolo della Libertà saremo al fianco del Governo, saremo al fianco dell'agricoltura italiana e, soprattutto, saremo al fianco degli agricoltori veri. Pertanto, noi del Popolo della Libertà voteremo «sì» a questo provvedimento.

con quello che provai a fare nel 1994-95 e non ho cambiato idea rispetto ad una situazione che non è assolutamente cambiata da quegli anni. Una situazione che era ricca di tante ombre, a partire dall'esistenza soltanto sulla carta - sottolineo, sulla carta - di soggetti inesistenti che aggravavano sempre di più la situazione dei veri produttori. Non mi pare che le attività di questi anni siano state rivolte a fare pulizia, veramente pulizia, e mi meraviglia che lei non l'abbia fatto preventivamente, signor

un decreto del genere, avrebbe inteso fare veramente pulizia delle cosiddette quote di carta delle tante cooperative inesistenti. i miei ricordi c'è anche il ricordo di un emendamento presentato ad un decreto particolarmente rigoroso, che il Governo dell'epoca presentò nel 1995. A tale decreto fu presentato un emendamento sull'autocertificazione. Io non so - o non voglio sapere o non posso sapere

da quell'autocertificazione in poi, cioè dalle ultime dodici campagne lattiere. Signor Ministro, con questo decreto avremmo preferito registrare qualcosa di più nuovo, di più moderno,

francamente non so proprio. Signor Ministro, questo è un provvedimento, come qualcuno di voi direbbe di altre misure, assistenziale e clientelare e per questo non intendo votarlo.

Ricorre domenica prossima, 8 marzo, come certamente sapete, la festa della donna. Non è, questa ricorrenza, solo un momento di rituale ricordo della rilevanza e della centralità della questione femminile nel nostro e negli altri Paesi. Certamente, c'è il ricordo e c'è la vicinanza affettuosa verso tutte le donne, quelle a noi più vicine negli affetti familiari, quelle che incontriamo negli ambienti di lavoro e nella vita sociale, quelle che nel nostro Paese e in tutto il mondo sono parte essenziale della società contemporanea. Oltre a questo ricordo, l'8 marzo deve però costituire per tutti, uomini e donne, un momento di riflessione e di verifica su quanto è stato fatto e su quanto resta da fare per assicurare una uguaglianza non soltanto formale (questa è già stata riconosciuta con lungimiranza dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale che, ed è significativo, sancisce l'uguaglianza "di sesso" come prima fra tutte le altre pur fondamentali uguaglianze), ma concreta ed effettiva. Ciò vale nel campo dell'istruzione, del lavoro, dei diritti familiari e in tutti gli altri campi che devono assicurare la tutela della dignità, della libertà e dell'eguaglianza femminile, a qualsiasi livello questa si manifesti. Episodi recenti di cronaca hanno portato nei mesi scorsi alla nostra attenzione il tema, purtroppo sempre attuale, della violenza contro le donne. forze politiche, Parlamento e Governo hanno già adottato misure significative e altre sono in corso di adozione con un consenso, spero, che possa essere il più ampio possibile. Ma, questa, è cosa che ci vedrà impegnati tutti i giorni. Oggi voglio solo ricordare e ringraziare, insieme a tutte le donne del nostro Paese, in particolare quelle che svolgono la loro preziosa attività nelle istituzioni, a cominciare dalla nostra. A loro va il mio ringraziamento e il mio saluto affettuoso e, consentitemi di anticiparlo, una sorpresa che, mi auguro, permetterà loro domenica prossima di poter meglio riconoscere l'affetto che il Senato, e la sua Presidenza, portano nei loro riguardi.

per il lavoro importante svolto sia in quella sede sia in Aula. Ringrazio tutti i colleghi che hanno dato vita a un dibattito interessante e utile per modificare, equilibrandolo ulteriormente, il testo che andiamo ad approvare.